È più o meno dal 2012 che proponete al Paese lo *slogan* che bisogna cancellare la riforma Fornero sulle pensioni e che bisogna avere un sistema tutto diverso. Anche gli ultimi mesi sono stati caratterizzati perennemente da questo *slogan*, che dà evidentemente per scontato che sia facile intervenire sul sistema previdenziale senza avere l'idea di dove portarlo. infatti di fronte al fatto che l'unica cosa che avete fatto è stata peggiorare una delle poche norme della legge Fornero che invece aveva trovato il gradimento delle lavoratrici; mi verrebbe da dire, visto che molti anni sono stati dedicati a migliorare il contesto e soprattutto a proteggere le condizioni più deboli. Non so se lo abbiate colto, ma il riferimento, ovviamente, è a opzione donna, che non è mai stata un favore alle lavoratrici, non lo è stata all'origine e non lo è tuttora nella norma, in quanto determinava una condizione di ricalcolo della loro pensione pur di pur di permetter loro di uscire anticipatamente; una delle poche forme, a differenza di altre che avete inventato negli anni, che non aveva grandi oneri per lo Stato. Eppure vi siete accaniti su questa: lo avete fatto l'anno scorso e con il disegno di legge di bilancio continuate a farlo. farlo. In verità credo che il problema sia che non capite la ragione per cui le lavoratrici sono disposte a perdere una parte della loro rendita pensionistica, pur di lasciare il lavoro prima. infatti a sfuggirvi l'idea che, finché non c'è una condivisione del lavoro di cura, finché non ci sono gli asili nido, finché non ci sono le strutture che permettano alle lavoratrici di affrontare contemporaneamente il lavoro e la condizione della loro famiglia, il loro lavoro varrà continuamente doppio e determinerà grandissima stanchezza. Ritengo pertanto che sarebbe bene che quest'Assemblea provasse ad ascoltare la domanda che ci viene dalle lavoratrici. Ognuno di voi, come la sottoscritta e come tanti altri, ha la posta inondata di domande di lavoratrici che chiedono

perché è un ciclo continuo, che inizia con le nascite e prosegue fino alla morte dei loro cari. Pertanto, da questo punto di vista, penso che davvero bisogni che ascoltiate quelle lavoratrici per oggi, per coloro che possono e vorrebbero ai criteri di opzione donna e la possibilità di avvalersene, ma anche rispetto ai discorsi che fate per il futuro. Non ci sarà un'occupazione femminile degna di questo nome e competitiva con il resto dell'Europa se non cominceremo a pensare che, se si fanno due lavori invece di uno e se ci si occupa della cura della famiglia e si sta contemporaneamente questo determina stanchezze e fragilità ben diverse da quelle maschili. Invece di continuare ad accanirsi su queste lavoratrici, forse sarebbe bene ripristinare quella norma e riconoscere loro che il lavoro di cura non è un fatto privato, che si svolge solo ed esclusivamente tra le mura di casa. Il lavoro di cura è ciò che ci permette di dire che abbiamo un *welfare* e le tutele.

sembrava che ci fosse una disponibilità a intervenire su questo. Alla Camera, in Commissione cultura, a giugno 2023 era stata approvata una risoluzione che riguardava proprio questo caso e intendeva risolvere il problema di centinaia di pensionati che si vedono liquidare la pensione,

che affronta alcune questioni relative alla previdenza. Molto spesso, in campagna elettorale ci si allarga molto nelle dichiarazioni, poi non sempre agli elettori e alle elettrici ritorna quello che alcuni promettono. Oggi siamo davanti a un caso molto più forte: non solo non ritornano le promesse (cancelliamo la Fornero), ma la maggioranza è riuscita in un intento che onestamente credevo impossibile per qualsiasi politico e cioè peggiorare di molto la legge Fornero. Questo è avvenuto per opzione donna, come ci ha ricordato la senatrice Camusso, e avverrà per i medici, per gli infermieri e per i lavoratori degli enti locali in modo drammatico, anche in termini generali:

volete fare tutto con ricalcolo contributivo, andando a far rimettere a ogni lavoratore e a ogni lavoratrice 300-400 euro al mese di pensione. È una vergogna, ma il massimo lo avete fatto

utile e degno il lavoro di quest'Assemblea e cerchiamo di lasciar svolgere gli interventi, da qualsiasi Gruppo provengano. Ovviamente passerò poi a chiamare nominalmente chi impedisce di svolgere i lavori. *(Brusio)*. Prego, senatrice Furlan,

che l'Ape sociale era stata pensata per i lavoratori e per le lavoratrici licenziati, per chi nella propria famiglia ha un figlio, un marito o una moglie con gravi problemi di salute cronici. *(Applausi)*. Era stata pensata per i lavoratori che ogni giorno svolgono mansioni usuranti, usuranti, spesso collegate a lavori pericolosi, in un Paese in cui ogni giorno abbiamo un bollettino di morti sul lavoro. Anche

come aventi diritto. Spero davvero, per il bene di tanti lavoratori e di tante lavoratrici, che sulla previdenza non facciate quello che avete promesso in campagna elettorale; almeno però non continuate a danneggiare

chiederebbero la possibilità di rientrare nei *benefit* che ci sono. È un fondo che non costa nulla allo Stato, perché sostanzialmente se lo pagano i lavoratori e le lavoratrici. Non si capisce perché

è costretto a portare in Aula un emendamento di questo tipo con la firma di un parlamentare, che interviene su scadenze già consolidate (perché quelle di cui stiamo parlando, per quello che riguarda la rottamazione-*quater*, sono previste al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre) 2023, per noi questo è un condono. Si sceglie con questo emendamento di abbandonare tutte le proposte che erano utili per i lavoratori e per le pensioni e la destra persevera con un vizio consolidato, quello di introdurre condoni al posto di misure utili per sostenere il lavoro e la crescita. *(Applausi)*. Riteniamo questo atteggiamento molto grave. Voglio tornare a chiedere al senatore Lotito di ritirare questo emendamento, perché per noi è la violazione di un principio chiaro: si interviene su scadenze già consolidate, configurando un vantaggio per gli evasori e uno svantaggio per chi le tasse le paga regolarmente.

lo Stato avrà una mancata entrata: questo è il dato fondamentale. Si adottano due pesi e due misure. Per questa ragione, insisto anch'io che venga ritirato, altrimenti voteremo contro.

all'esigenza di consolidare qualcosa che l'Agenzia delle entrate già fa, non si riaprono termini post-votazione dell'emendamento. Si faccia una riformulazione che

ciò che non può Giorgia Meloni, ciò che non può Matteo Salvini e ciò che non può nessun altro degli esponenti della destra di questo Paese può il senatore Lotito. Il senatore Lotito è il vero capo della maggioranza, colleghi, dobbiamo dargliene atto e dobbiamo in qualche modo anche rendergli onore in quest'Aula. Vedete, in Commissione questo provvedimento è stato presentato dal sottosegretario Freni, da tutti gli esponenti del Governo, dal ministro Ciriani come a saldo zero:

in un modo indecente da un Governo che non vuole prendere atto che la sanità è al collasso e alcune persone sono penalizzate sotto il profilo pensionistico, come infermieri e come medici che hanno fatto la loro parte rischiando la loro vita durante l'emergenza Covid. *(Applausi)*. No, tutto questo non si poteva fare; ma naturalmente, per essere coerenti e sdraiati sulle esigenze del senatore Lotito, si può rendere questo decreto-legge da saldi invariati a saldi molto variati. Complimenti, avete eletto il vostro nuovo *leader* della maggioranza e ne prendiamo atto. Credo che i cittadini abbiano molto da ridire circa il fatto che si diano priorità a queste cose anziché agli infermieri e ai medici di questo Paese. Buon lavoro al Governo e buon lavoro al

sui corretti binari. Mi rivolgo a lei, Presidente, perché ho sentito terminologie completamente sbagliate e fuorvianti. Riportiamo il dibattito sull'emendamento, che ha il parere favorevole perché è un emendamento di tecnica di bilancio. Noi chiudiamo la contabilità precisamente il 18 dicembre e, quindi, con una scadenza ancora possibile e in corso,

soldi nelle casse dello Stato. I termini è giusto utilizzarli, ma questo non è un condono; si tratta soltanto di un aggiustamento di contabilità di bilancio.

l'invito che faccio è che tutto questo entusiasmo e questa visibilità che date al senatore Lotito rischia di diventare per lui un motivo di vanto. Quindi, anziché fare opposizione, rischiate di fargli un favore, se continuate a dire che lui può quello che tanti altri non possono. L'invito che rivolgo è: usate con attenzione il vostro metodo di fare opposizione. Così come, se vogliamo in qualche modo far sì che la classe politica ritrovi un po' di credibilità, impariamo a chiamare le cose per quello che sono: questa è una rimessione in termini. C'è lo spostamento di un termine per il versamento delle due rate. Lo dico al senatore Manca, che segue le questioni in Commissione bilancio e quindi dovrebbe conoscere bene la materia.

sapete che questa Presidenza è sempre molto attenta al linguaggio.

sul metodo, sulle questioni politiche, sulle polemiche, come maggioranza siamo sempre disponibili a comprendere e anche ad ammettere se c'è qualche questione che bisogna migliorare, facendo anche, qualche volta, autocritica. Evitiamo però che ne derivi una lotta nell'Aula, perché l'intento era assolutamente un altro. Ad ogni modo, chiamiamo le cose con il loro nome: non è un condono, è una rimessione in termini. Per questo voteremo a favore

io credo che non si possa far passare sotto silenzio quello che è accaduto.

Presidente, l'emendamento 5.0.19 fa parte di un pacchetto di emendamenti che abbiamo presentato come Gruppo e che sono stati tutti respinti dal Governo. Il tema riguarda i mutui, in particolare quelli a tasso variabile e il sostegno alle famiglie e alle imprese. Abbiamo presentato diversi emendamenti su questo e viene da sorridere pensando solo che qualche mese fa, per esempio il 29 giugno, «Il Sole 24 Ore» titolava: «Meloni al Consiglio europeo: sui mutui dobbiamo fare di più»;

la tassa sugli extra profitti servirà per aiutare le famiglie sui mutui». Se fate una ricerca su Google sulle parole «mutui« e «Governo Meloni» vengono fuori tantissime parole, inversamente proporzionali alle risorse e alle misure concrete che avete predisposto per le famiglie e le imprese su questo tema. Voi sapete che il livello dei tassi di interesse, a causa della congiuntura macroeconomica, è particolarmente cresciuto in questo Paese. Noi abbiamo individuato una serie di pacchetti,

Ebbene, il Governo ripetutamente ha detto di no. È giusto che gli italiani sappiano. Quei milioni di famiglie e di imprese che hanno visto crescere in modo repentino il costo del proprio finanziamento per investimenti e per mutui per abitazioni e per la prima casa, non c'è stata la possibilità di inserire e di far nascere, come dicono i nostri emendamenti, due fondi di sostegno che sarebbero serviti ad aiutare esattamente famiglie e imprese. questo è un momento fondamentale nel quale, se erodiamo la capacità di spesa degli italiani in ragione del maggior costo dell'indebitamento, (questo riguarda sia le imprese che le famiglie) ciò si traduce in una riduzione della domanda che va a incidere in modo ancora più significativo sulle aspettative di crescita del prodotto interno lordo. Un prodotto interno lordo che, nella legge di bilancio, voi prevedete che crescerà per cento, quando tutti gli organismi internazionali danno lo 0,7 per cento, peraltro allineato anche a quella che è la dinamica europea. Ecco, in questo contesto e con questa misura era necessario dare un segnale. Le risorse erano coperte. In ogni caso, ci sarebbe anche quella tassa sugli extraprofitti che avete cancellato. Fa riflettere che, rispetto a tutte le risorse che fino agli ultimi giorni sono state messe sul tavolo da questo Governo per una serie di misure del tutto irrisorie, frammentarie, non si sia trovato, da parte del Governo, ma soprattutto da parte dei colleghi della maggioranza che so essere sensibili a questi temi, il coraggio di dire sì ad un emendamento che non riguarda la destra o la sinistra, ma riguarda le famiglie degli italiani e un momento particolare del nostro equilibrio socio economico. Quindi, da questo punto di vista, il parere del Governo e della maggioranza diventa una responsabilità pesante che iniziate a caricarvi sulle vostre spalle.

che rispondano ad esigenze mediche non soddisfatte. Detto così, è ovvio che non sia particolarmente chiaro, se non agli addetti ai lavori, di che cosa esso tratti. Per fare un esempio concreto in modo che tutti possano comprenderne le esigenze, si tratta delle macchine di perfusione che si utilizzano nei casi di trapianto d'organo. Queste macchine consentono di utilizzare che, ad oggi, senza la loro disponibilità, andrebbero persi, perché non utilizzabili. Consente anche di allungare i tempi di trasporto degli organi dal luogo di prelievo al luogo di impianto. Consentono anche, a volte, ai medici di avere tempi di intervento più adeguati a conciliare ore di riposo in modo che abbiano una prontezza maggiore nel momento in cui effettuano gli interventi.

ordine del giorno e mi auguro che la maggioranza voglia fare una riflessione su questo tema, perché è davvero fondamentale per la vita delle persone.

la disponibilità a esprimere un parere favorevole, aggiungendo la mia firma e quella della senatrice Murelli, perché entrambi abbiamo partecipato a un convegno insieme con la senatrice Pirro, che è anche presidente dell'intergruppo

vorreisostenere questo importante ordine del giorno, aggiungendo la firma di tutto il Gruppo Italia Viva, augurandoci però che queste risorse possano individuarsi già nella legge di bilancio, perché sarebbe un grande segnale. Abbiamo lavorato in modo trasversale, come ha detto anche il collega Romeo, con tutti i colleghi e le colleghe della Commissione, quindi l'auspicio è che si possa davvero - e lo chiedo al Governo - non solo esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G5.0.300, ma soprattutto trovare le risorse nella legge di bilancio.

sul tema della sanità. Abbiamo ancora un problema enorme che è l'articolo 33. C'è tempo per cancellarlo ed evitare il taglio delle pensioni di medici, infermieri e personale della scuola. Mi auguro che la legge di bilancio sia veramente l'occasione per evitare quello che sarebbe un nuovo caso esodati. Leggiamo sui giornali che su questo punto c'è un'apertura del ministro Schillaci, ma non è sufficiente: quell'articolo va semplicemente cancellato. chiedere di sottoscrivere come Capogruppo in Commissione affari sociali e sanità questo ordine del giorno. Ringrazio la collega Pirro per la sua sensibilità e intelligenza

Signor Presidente, il parere è favorevole; il Governo accoglie certamente l'indicazione dell'Assemblea, ovviamente compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ma è chiaro che ci sarà la massima attenzione per poter reperire le risorse che sono destinate alla sicurezza e alla salute dei nostri cittadini.

Sulle banche noi andiamo dritti. Nei primi sei mesi hanno fatto più di 20 miliardi di utili, quindi a fine anno ci saranno 40 miliardi di utili delle banche italiane senza che però nemmeno una parte di questi utili tornino ai risparmiatori che hanno soldi sui conti correnti». *(Applausi)*. È vergognoso! Noi andiamo dritti. Una piccola parte potremmo usarla per aumentare pensioni e stipendi dei lavoratori italiani; Se a fine anno le banche italiane invece di guadagnare 40 miliardi, ne guadagnassero 30 o 35, i loro azionisti saranno comunque contenti. *(Applausi)*. Con questi soldi aiuteremo, perché indietro non si torna, tanti lavoratori. Matteo Salvini, 28 agosto 2023.

Siccome sulla norma extraprofitti indietro non si torna, noi presentiamo un emendamento che propone di far sì che quella tassa funzioni veramente,

fiscale legato all'andamento dei prezzi del carburante. È di tutta evidenza che, a seguito dell'impennata, avvenuta in particolare nei mesi scorsi, dei prezzi della benzina e, più in generale, dei carburanti, il Governo, o meglio lo Stato, attraverso il meccanismo automatico di applicazione delle accise ha avuto un aumento di gettito. quindi, anche per mantenersi coerenti rispetto alle cose che sono state dette, che si debba introdurre comunque un meccanismo di blocco delle accise una volta che si raggiunge il *plafond* stabilito all'interno della legge di bilancio. Invece qui cosa succede? Avviene che, se fatto 100 in legge di bilancio il gettito delle accise e e il valore del carburante aumenta, lo Stato continua ad incassare e quindi c'è una doppia penalizzazione nei confronti dell'utenza e dei cittadini. Quindi, noi ci troviamo ad avere una classe politica che a parole dice che bisogna bloccare l'aumento del prezzo del carburante e nei fatti lascia correre che lo Stato, di fatto, faccia il biscazziere su un andamento da cui le casse dell'Erario hanno un ritorno positivo. Questo secondo elemento, dal nostro punto di vista, non è accettabile. Quindi, per essere coerenti con le cose che si sono ripetutamente dette, anche a livello governativo, occorrerebbe votare a favore di questo emendamento.

7.301 riguarda un tema molto delicato, perché - com'è noto - a legislazione vigente dal prossimo gennaio per il gas e da aprile per la luce finirà il regime di maggior tutela e 5 milioni di famiglie andranno in libero mercato. È un passaggio molto delicato che avviene in una fase complessa. Nel 2022 abbiamo avuto la peggiore crisi energetica da cinquant'anni, che ha portato ad un'impennata dei prezzi della luce del gas e ad un'estrema volatilità dei mercati, mentre il 2023 è un anno purtroppo segnato da una guerra drammatica in Medio Oriente e da mercati ancora lontani da una condizione di normalità. Invito i colleghi a guardare il monitoraggio che ARERA fa delle offerte di libero mercato disponibili: a novembre la media delle offerte per un utente tipo della luce a libero mercato ha prezzi superiori del 17 per cento rispetto alla tutela. Il differenziale è addirittura del 21,4 per cento per il gas (mercato libero rispetto al regime di tutela). Questi 5 milioni di famiglie non sono state informate a dovere, sono in una situazione di grande incertezza, vengono bombardate da campagne di *marketing* aggressive e le state esponendo ad una vera ad una vera e propria stangata, dopo due anni di inflazione che ha eroso il potere d'acquisto dei redditi. Il rinvio era stato ipotizzato più volte dal ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ed è oggi purtroppo scomparso dai radar del Governo. In compenso, due giorni fa, il Consiglio dei ministri ha annunciato una campagna di comunicazione, a trenta giorni dall'avvio del libero mercato per il gas. Si fa una campagna di comunicazione che andava promossa mesi e mesi fa per rendere gli utenti consapevoli. Qui il tema non è una campagna di informazione a babbo morto, ma è il rinvio che voi stessi avete ipotizzato per preparare al meglio questo passaggio che è stato deciso anni fa, ma in una fase completamente diversa, quando non c'era la crisi energetica che ci ha investito e non c'era questa volatilità dei prezzi. L'emendamento che sto illustrando non per mettere in discussione questo passaggio, ma per prepararlo al meglio a difesa di questi cinque milioni di famiglie.

facciamo ancora largamente uso e dai quali, così come dagli extraprofitti, sarebbe possibile dedurre almeno 20 miliardi. Si otterrebbero in tal modo due benefici: maggiori entrate per le casse dello Stato e e minori immissioni inquinanti nell'aria e, quindi, minore inquinamento. Sarebbero benefici rispetto alla crisi climatica che stiamo vivendo. Questo emendamento è il primo, ma ce ne sono almeno altri due che vanno nella stessa direzione. Come MoVimento 5 Stelle chiediamo a quest'Assemblea un supplemento di riflessione rispetto a questo indirizzo e rispetto al parere sull'emendamento 7.0.3 perché possa essere approvato, così come ci chiedono

alcune proroghe nell'attuazione del superbonus 110 per cento, misura che evidentemente è ben vista da parte almeno di un pezzo della maggioranza e che - a mio avviso - va sostenuta. Chiederei dunque a tutte le forze di opposizione di aiutare e sostenere l'emendamento presentato da una forza di maggioranza che forse ha qualche problema con gli alleati. Noi siamo sempre disponibili a dare una mano e anche mettere il dito in qualche piaga. *(Applausi)*.

invito al ritiro. Presidente, noi ci rimettiamo alla decisione del Governo. Evidentemente ci sono delle questioni tecniche. Auspichiamo però che in futuro si possa riconsiderare questo aspetto. Abbiamo sanato un'ingiustizia che durava da anni, per quanto riguarda gli aspetti contabili. Speriamo che anche gli altri professionisti, i consulenti del lavoro, possano accedere alla presentazione telematica

che riguarda una serie di proposte che con i senatori Franceschelli e Zambito, a nome di tutto il Gruppo PD, abbiamo avanzato affinché vi fosse una risposta all'alluvione che ha colpito la Toscana il 2 novembre. Come è ben noto a tutto l'Emiciclo, il 2 novembre si è abbattuto un nubifragio sulle parti centrali della nostra Regione. Ci sono stati otto morti otto morti e danni per 3 miliardi di euro. Vi era la grandissima necessità che il Governo desse immediatamente delle risposte concrete e adeguate.

lo svolgimento di tutte le azioni necessarie. Ci duole constatare che in Commissione questo emendamento è stato quasi completamente ignorato e respinto. Io vorrei che fosse chiaro che questo Governo, che è così celere e rapido quando si tratta di mettersi sull'attenti di fronte alle richieste del senatore Lotito, *(Applausi)* è poi molto lento e incapace di dare qualsiasi risposta quando si tratta di rispondere ai bisogni di una Regione colpita da un'alluvione che ha causato otto morti e tre miliardi di danni. Quindi, il mio intervento è anche una richiesta al Governo affinché di perseguire una linea di opposizione vergognosa a una richiesta sacrosanta. Sapete fino ad oggi, di fronte a tre miliardi di danni, quanto ha stanziato il Governo per la Toscana? milioni. Si tratta - basta usare una calcolatrice - dello 0,2 per cento del fabbisogno. Non c'è di fronte a noi né un decreto-legge, né una bozza di decreto-legge che metta delle risorse adeguate. Non ci sono impegni concreti per lo stanziamento di fondi che servano perlomeno a contrastare le emergenze più gravi. In compenso, in questo decreto-legge è stata inserita una proroga canzonatoria dei termini per il versamento di contributi e tributi: proroga di pochissimi giorni che è suonata come un pugno in faccia, uno schiaffo alle tante imprese che hanno subito danni immensi a causa dell'alluvione. Smettete di prendere in giro i toscani. Smettete di prendere in giro le aziende, le imprese, gli enti locali, le famiglie della Toscana. Date delle risposte. L'accoglimento di questo emendamento sarebbe una prima occasione per dare risposte. Io credo che chi sceglierà di votare contro questo emendamento si assumerà una responsabilità molto grave e metterà la faccia su una decisione sbagliata, vergognosa, indecorosa, soprattutto alla luce del fatto che che si è pronti a fare spazio a richieste sbagliate e si chiude la porta in faccia alle richieste giuste. Questo non va assolutamente bene.

Signor Presidente, mi spiace ovviamente perché il tema è sentito da tutti, ma tecnicamente è impossibile inserire una specie di disegno di legge aggiuntivo in questo decreto. Esprimo quindi parere contrario

Presidente, il Governo si è dimenticato di un po' di cose in questo provvedimento, che doveva essere non oneroso, ma che poi lo è diventato; cose che incidono sulla carne viva dei cittadini, tra cui il tema degli affitti, della casa, del diritto dell'alloggio e, in questo senso, il tema ancora più grande del diritto allo studio. Il diritto allo studio, nel nostro Paese, ancora oggi non è pienamente realizzato in tutte le sue forme, nonostante ci riempiamo la bocca, in quest'Aula, dei temi riguardanti i bambini i bambini e il loro futuro, le diseguaglianze, l'investimento sul capitale umano. In questo emendamento noi affrontiamo la grande questione del trasporto scolastico. Signor Presidente, studiare Costa circa 1.800 euro l'anno in età scolastica a famiglia, e questo costo differisce da Regione a Regione, creando delle ingiustizie e diseguaglianze che arrivano fino a mille euro

costa 5,43 euro al Sud, che diventano 7,40 nel Centro Italia. Sui trasporti ferroviari, ci sono Regioni virtuose come l'Emilia-Romagna, l'Umbria, il Lazio, la Campania e la Provincia autonoma di Trento, dove l'abbonamento annuale è molto conveniente e vede integrato anche il trasporto pubblico urbano. Le peggiori sono, invece, il Piemonte, la Lombardia e la Sicilia, con una differenza annuale di oltre mille euro. In questo emendamento e negli altri che seguiranno noi abbiamo presentato delle risposte,

beneficiari sono 4.974: 4.974 bambini e ragazzi meriterebbero una borsa di studio, le cui famiglie dovrebbero essere aiutate dallo Stato e non hanno accesso a tali fondi. È un'ingiustizia.

questo emendamento prevede un aumento da sei milioni a dieci milioni per il fondo affitti degli studenti. studenti. Un Paese che non guarda al futuro non guarda ai propri studenti. Ed è un Paese sordo anche alla richiesta, alla voce che hanno alzato gli studenti, con le tende nelle piazze. non capisce quanto oggi sia ancora più difficoltoso, anche per le famiglie che vivono l'inflazione, investire sui propri ragazzi. Questo Paese si deve prendere cura allo studio deve essere effettivo; un Paese che non guarda al futuro, non guarda ai propri studenti. Su questo noi chiediamo che anche la maggioranza si renda conto di cosa significa oggi ancora di più il costo da una famiglia per uno studente universitario. Oggi il costo degli affitti è pari a quasi 350 euro al mese,

permetterci di essere sordi al richiamo chiaro che hanno fatto gli studenti e le studentesse. Oggi solo il 28,3 per cento della popolazione tra i venticinque e i trentaquattro anni riesce a conseguire un titolo universitario; il tasso di abbandono è cresciuto

quello che sto per pronunciare non è solo un intervento con il quale sostengo le ragioni di un emendamento, ma vuole essere, tramite la Presidente, anche un appello ai colleghi della maggioranza rispetto alla vicenda delicatissima e urgentissima che riguarda l'ex Ilva. E questo appello voglio rivolgerlo a tutti voi, perché sono certo possiate capire cosa sta accadendo e intervenire per cambiare direzione di marcia. Se così non farete, vi assumerete davvero una grande responsabilità. Cosa deve accadere, infatti, cari colleghi, affinché voi possiate capire che, con quello che sta avvenendo, si sta compromettendo il futuro della siderurgia italiana, il futuro di 10.500 lavoratori, di altrettanti lavoratori dell'indotto, degli stabilimenti di Taranto, di Genova e di Novi Ligure? Cosa deve accadere ancora, colleghi, per capire che ieri l'assemblea dei soci non ha prodotto nulla ed è stata rinviata ancora la decisione al 22 dicembre, cioè a Natale, tanto dei lavoratori che non sanno come passeranno il Natale chi se ne importa? Cosa deve accadere ancora, colleghi, perché voi vi rendiate conto che le sigle sindacali hanno indetto quarantott'ore di sciopero per evitare che si chiuda l'altoforno, così come forse vorrebbe l'azienda, per interrompere le produzioni? Cosa deve accadere ancora perché vi rendiate conto che c'è un socio privato che probabilmente non ha alcun interesse a investire in Europa, anzi, che forse trova vantaggioso eliminare dal mercato europeo un proprio *competitor*? E parlo

tutto questo sta avvenendo nel silenzio, nell'afasia, nella grave responsabilità del Governo. Ricordate, colleghi, che con un decreto si è stabilito che c'erano 680 milioni per procedere in una certa direzione e sono stati bruciati per pagare le bollette. C'era un miliardo per il piano di decarbonizzazione collegato al PNNR è stato tolto di mezzo. E poi il ministro Fitto ha firmato un *memorandum* *motu proprio* di cui non conosciamo i contenuti, che in quest'Aula abbiamo chiesto più volte di conoscere. Non si sa nulla. Non si capisce come possa andare avanti e questo - guardate non è proprio possibile. Non ce lo aspettavamo dal Governo che voi chiamate "della Nazione".

fatelo prima del 22 dicembre; approviamo questo emendamento, con il quale cambiamo la *governance*; attiviamo un aumento di capitale del socio pubblico rappresentato da Invitalia e lo attiviamo subito

che fino ad oggi è stato all'oscuro di tutto, e anche una parte del Governo, se non sbaglio, le parti sociali, le associazioni di categoria, quelle parti della siderurgia italiana che possono concorrere a un nuovo progetto per dare una prospettiva a

l'emendamento 13.21, con il qualecerchiamo di offrire supporto alle imprese del settore ceramico, che sono tra quelle che hanno subito maggiormente le conseguenze del caro energia raddoppiando le quote di remunerazione del servizio di interrompibilità. Sarebbe un bel segnale per rispondere a una forte, sentita, grave richiesta d'aiuto che proviene appunto dal settore ceramico.

e un coordinatore della Protezione civile sono stati sanzionati, anche poi con conseguenze penali, a seguito di un tragico incidente che ha coinvolto un volontario. L'emendamento che è stato introdotto dal Governo introdotto dal Governo chiarisce quali siano effettivamente le responsabilità dei volontari della Protezione civile, mettendo in sicurezza la loro attività che è estremamente importante. Voglio ricordare che in Italia ci sono un 1.300.000 volontari della Protezione civile.

di spopolamento e della necessità di favorire i giovani e le donne, si chiede di aumentare di 10 milioni il fondo e si dice di no? Siamo davvero in una situazione nella quale

sono costretti a lavorare in agricoltura sono i sottopagati, i clandestini, quelli che in sostanza facciamo finta di non vedere. E non promuoviamo invece l'attività dei giovani e delle donne. Vorrei sottolineare questo dato e

il Governo deve evidenziare che la proposta presenta profili di criticità, in quanto inciderebbe su contenziosi in atto ed è suscettibile di generarne ulteriori, atteso che attiene ad annualità di fondi già ripartiti. Pertanto, su questo emendamento il Governo si rimette all'Assemblea.

siamo di fronte a una situazione di grande difficoltà. Ve lo dico perché ho avuto l'occasione di sentire con le mie orecchie il prefetto di Genova

Lo dico per primo, avendo fatto il Ministro dello sviluppo economico in una stagione complicata, e mi assumo una parte delle responsabilità di ciò che ancora non si è risolto in quello stabilimento. Ho maturato però una certezza sola, che non sarà una gestione di mercato e privata a poter garantire l'occupazione, la reambientalizzazione e la decarbonizzazione di quel sito.

le risorse e il percorso di decarbonizzazione necessari allo stabilimento di Taranto a tutela dell'occupazione e soprattutto della vita delle persone che vivono in quel territorio. Perdere questa occasione e tornare invece a sperare che ci sia un imprenditore dell'acciaio che investa in uno stabilimento come quello, con le necessità e le e le difficoltà che ha e con la concorrenza che nella produzione di acciaio arriva da Paesi molto lontani da noi, dove le tutele ambientali e dei diritti di lavoratori e i costi delle materie prime sono totalmente diversi da quelli che abbiamo nel nostro Paese, è follia e utopia. Non perdiamo l'occasione, non retrocediamo da un impegno preso, che è quello di aumentare la presenza dello Stato nel capitale sociale di quello stabilimento. Individuiamo i *manager* migliori per gestirlo, ma facciamo sì che la linea e

hanno presentato emendamenti a favore dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile nel settore agricolo. Noi, come Gruppo, voteremo favorevolmente a tutti gli emendamenti che vanno in tale direzione, ricordando che questa settimana l'Ispettorato nazionale del lavoro ha certificato ben 44.000 dimissioni volontarie di donne a seguito della nascita del primo o del secondo figlio. Questo significa che lo Stato, quindi noi, attraverso la nostra attività legislativa, dobbiamo sostenere maggiormente in tutte le forme l'occupazione femminile, sia nel lavoro dipendente, sia nel lavoro autonomo e imprenditoriale. L'occasione per cominciare a dare un segnale sarebbe il voto unanime dell'Assemblea su questi emendamenti.

comuni interessati dalla tratta autostradale A24 e A25 di interloquire con il Ministero, con il gestore dell'autostrada (oggi ANAS, prossimamente Strada dei parchi)

la tariffa di tale tratte autostradali è tra le più care d'Europa. Andando avanti nei successivi emendamenti, e in linea con quello che ho appena riferito su una tariffazione così alta, quello che chiedo non è altro che ciò che è sempre stato chiesto da tutti i Gruppi politici quando si parlava di A24 e A25, ovvero di prevedere una formula di riduzione delle tariffe per coloro che, per forza di cose - lo sottolineo - devono utilizzare l'autostrada per potersi spostare. Più precisamente, parlo dei pendolari che provengono dall'Abruzzo per recarsi a Roma (città capitale) per questioni di lavoro, di chi si sposta per motivi sanitari e per curarsi o dei giovani studenti, già soggetti a un caro affitti indescrivibile. Chiedo quindi di portare un'attenzione particolare a queste persone

si è astenuto sull'emendamento del Governo, presentato per mano dei relatori, che prevede la riconsegna della gestione delle autostrade A24 e A25 da ANAS

i membri del Governo stesso, in altre circostanze, in altri sedi, hanno egualmente proposto. Sono quindi certa che il Governo avrà un'attenzione particolare per questi temi.

quello che è scritto qui corrisponde esattamente a quanto dichiarò l'onorevole Francesco Lollobrigida prima di andare al Governo, cioè prima di diventare Ministro e, incidentalmente, anche capostazione.

Signora Presidente, torno a ricordare - visto che sono passati alcuni minuti - che questo Governo dice di no al sostegno ai mutui degli italiani. al tema delle imprese; con questo emendamento ci rivolgiamo alle famiglie, con un costo che è davvero sostenibile, perché cumula massimo 250 più 50 milioni

vi sono dei sottocasi, quindi parliamo di un numero di cittadini che si può gestire. Noi proponiamo una misura di credito d'imposta per la parte eccedente del costo del mutuo,

per dare la possibilità, a coloro che hanno visto aumentare questi mutui, ma anche a coloro che ne hanno chiesto la rinegoziazione o che hanno adottato altre misure, come l'allungamento della rateizzazione, di avere un incremento del reddito disponibile e quindi di tornare a

dagli italiani. Questo Governo insiste molto sul credito d'imposta, per alcune questioni, ed è molto attento ad alcuni settori. Qui si fa riferimento a tutti gli italiani; magari questi italiani non sono sportivi, non sono giocatori di calcio, non sono soggetti attenzionati da alcuni interessi, ma in questo momento chiedono semplicemente un sostegno aggiuntivo a questo Governo e a questa maggioranza,

Signor Presidente, in poche parole, il nostro Paese è in ritardo nell'approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Tutte le volte che discutiamo in quest'Aula di alluvioni, di eventi climatici estremi, di disastri e di ristori a cittadini e imprese ci occupiamo dell'emergenza e non ci occupiamo mai della prevenzione e della pianificazione. *(Applausi)*. Siamo in ritardo e chiediamo che tale Piano sia attuato. Un atteggiamento positivo in questo senso, che peraltro naturalmente è neutro, perché poi andiamo a scriverlo il Piano, a scriverlo il Piano, è anche la migliore risposta al rischio che anche in questo nostro Paese, tra le fila di quelli che lo rappresentano, ci siano negazionisti o persone che minimizzano le problematiche legate al caos climatico.

di cui in premessa sulle politiche tariffarie adottate a tutela dei fruitori dell'infrastruttura».

tra gentiluomini e gentildonne di non fare polemica su questo argomento. C'è stata una deriva ideologica, che ha un nome e un cognome, da parte di alcune forze politiche che hanno messo in discussione un tema, quello dell'A24 e dell'A25, tanto sulla gestione, quanto

perso due volte in ambito giudiziario e siamo stati condannati a spese che potevano essere di 3, 4 o 5 miliardi di euro. Questa transazione non soltanto mette una parola fine alla

sbadata a livello amministrativo, su un'onda emotiva che non deve condizionare gli uffici e i Ministeri. Ricordiamo chi stava festeggiando con spumante o *champagne* (non ricordo esattamente sotto Palazzo Chigi, quando ci fu la statalizzazione delle autostrade, salvo poi oggi aver cambiato idea. Il tavolo di cui si parla da anni. Io ne ho fatto parte negli ultimi cinque o sei anni ed ho sempre partecipato. Il ministro Salvini e il vice ministro Bignami non hanno alcuna intenzione di far venir meno l'interlocuzione con i sindaci, tanto è vero che hanno continuato ad incontrarli e continueranno ad incontrarli ancora in futuro, con noi che faremo parte di quel tavolo e che li assisteremo. I sindaci continueranno ad essere protagonisti. Pertanto, chiedo anche al Governo, nella riformulazione dell'ordine

non tanto per la famiglia Toto, dei cui interessi non devo occuparmi io, ma per i 1.700 dipendenti che, per colpa di qualcuno che, a livello ideologico, ha portato avanti una battaglia sconnessa

lo ha affrontato, lo ha risolto e oggi siamo a festeggiare il fatto che 1.700 persone passeranno il Natale in santa pace. Questa è la vittoria dello Stato!

emendamento del Governo, depositato per mano dei relatori, è stato soppresso: a normativa vigente, è soppresso. Mi chiedono, cioè, di riformulare un testo in maniera scorretta. Chiaramente, non lo accetto e ricordo nuovamente a quest'Assemblea e, prima di tutti, a me stessa

nella seduta del 3 agosto 2022, n. 737, tal quale approvato ed accolto dal Governo Draghi. Ora, qui, voi state negando ciò che a voi è stato concesso. Voi prima pensavate di fare qualcosa e ora ci state ripensando,

di andare a beneficiare il territorio in questo dibattito sulll'interlocuzione con i sindaci; c'è la volontà di spostare l'attenzione rispetto a una soluzione della problematica che è stata trovata da questo Governo e non da quelli precedenti (alcuni dei quali lo hanno creato), per la quale molti hanno festeggiato. *(Applausi)*. Noi abbiamo risolto questo problema, abbiamo portato a casa la soluzione; non hanno votato contro in Commissione, perché hanno riconosciuto che siamo stati bravi, e adesso si va a guardare il dito e non la luna, si va a parlare nell'interlocuzione con i sindaci. Guardo i colleghi della Lega, guardo il mio amico Massimiliano Romeo e guardo negli occhi anche tutto il resto del centrodestra: non esiste il fatto che in futuro manchi l'interlocuzione con i sindaci del territorio. Il tavolo c'è, ci sarà e il ministro Salvini, così come il vice ministro Bignami, continueranno a portare avanti un'interlocuzione che negli ultimi dieci anni è stata portata avanti proprio per risolvere le problematiche create dai Governi che oggi non ci sono più per scelta degli italiani.

Colleghi, se c'è uno spunto polemico in una dichiarazione di voto è evidente che poi viene raccolto

Signora Presidente, lo so che la verità fa male, non mi vogliono far continuare. Noi abbiamo ottenuto anche il blocco dei costi dei pedaggi al 2017. Questo significa che... Senatrice Di Girolamo, adesso questo diventa un richiamo formale, per cortesia. Lei ha già fatto la sua esposizione con la *vis* polemica che ha ritenuto necessaria, adesso consentiamo al senatore Liris di proseguire.

*(FdI)*. Nella transazione tombale di 500 milioni, rispetto agli svariati miliardi che avremmo dovuto dare alla famiglia Toto, abbiamo chiesto il blocco delle tariffe dei pedaggi al 2017,

cui tanti costi dei pedaggi in altre autostrade vanno aumentando. Apriremo una trattativa con il gestore per quanto riguarda i pendolari, chiaramente avranno un trattamento diverso proprio per la fruizione costante dello stesso tratto di strada. Su questa pagina, dunque, anche in Commissione mi sono comportato in una certa maniera. Avevamo detto che non doveva essere elemento di confusione, ma sta diventando un momento per andare a guardare il dito e non la luna rispetto a un'interlocuzione con i sindaci che non è mai mancata da parte del centrodestra per salvare il territorio rispetto alle scelte dissennate di chi oggi strilla dalla parte della minoranza e che continuerà a maggior ragione oggi che siamo in maggioranza e al Governo.

Fratelli d'Italia chiede agevolazioni tariffarie per i pendolari delle A24 e A25. Non sono sufficienti azioni tampone per risolvere le criticità di un'arteria autostradale che tocca 113 Comuni di Lazio e Abruzzo. Servono interventi strategici per ridare dignità a quelle popolazioni che vivono in aree in cui le infrastrutture sono carenti. Non è accettabile che in Italia ci siano delle zone dove si viaggia gratuitamente, come previsto per la A22 per gli abitanti di Bolzano, grazie a Fratelli d'Italia, così come in passato per molte altre occasioni, e altre nelle quali i cittadini sono costretti a pagare cifre esorbitanti per muoversi, mentre i concessionari incassano, come nel caso della Strada dei parchi, circa 180 milioni di euro dai pedaggi. Fratelli d'Italia è sempre stato attento a queste problematiche e, dopo aver partecipato con i sindaci ai presidi presso i caselli autostradali, oggi ha incontrato nuovamente gli stessi amministratori locali per dare loro sostegno e per chiedere al Governo di prevedere per i residenti di quelle aree di percorrere gratuitamente

Mi stupisce il parere contrario anche dopo la trasformazione in ordine del giorno quando in Commissione, in realtà, alcuni pareri dei Ministeri competenti erano parzialmente favorevoli e quelli contrari erano dovuti al fatto che era necessario un chiarimento sulla platea di cui stiamo parlando. Vorrei chiarire a tutti di cosa parliamo. Parliamo di atleti di rilievo nazionale che, ad oggi, non vengono arruolati nelle Forze dell'ordine e nella Polizia di Stato perché affetti da difetti del metabolismo glucidico o lipidico. Stiamo parlando generalmente di diabete di tipo 1 e iperlipidemie familiari; cose che non confliggono con la vita quotidiana, tanto che questi atleti arrivano anche a svolgere competizioni internazionali. ci possa essere una riflessione su questi aspetti e magari un impegno a "valutare l'opportunità di" invece che una bocciatura in questi termini anche perché è davvero anacronistico che ancora venga impedito il loro arruolamento. In ogni caso sarà mia cura cercare di interloquire con i Ministeri competenti per far capire di cosa parliamo e soprattutto dei dei numeri irrisori di cui stiamo parlando.

perché con questa proposta abbiamo inteso ripristinare le risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità. Il Fondo conteneva 100 milioni che questo Governo ha pensato di tagliare. Abbiamo pensato anche di rifondere il Fondo per il sostegno al ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare per 70 milioni, che questo Governo ha deciso di tagliare, e di aumentare quello per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di 8 milioni per l'anno 2024 e 2 milioni per l'anno 2025.

aveva promesso che si sarebbe occupata di attuare la legge delega per l'implementazione del progetto di vita delle persone disabili e di migliorare l'*iter* di accertamento dell'invalidità civile. Aveva proposto un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e aveva promesso modifiche alla legge sul dopo di noi. Aveva anche promesso interventi per la vita autonoma autonoma delle persone con disabilità e anche che si sarebbe occupata del riconoscimento del *caregiver* familiare. Dopo un anno e due mesi non abbiamo visto ancora nessuna proposta del ministro Locatelli e invece vediamo questi tagli. Si vedono tagliare le risorse di fondi estremamente importanti. Siccome, Presidente, non basta istituire un Ministero per dare le risposte che attendono le persone con disabilità, i loro familiari e i loro *caregiver*, penso che sarebbe opportuno che tutta l'Aula appoggiasse e sostenesse questo emendamento, in quanto propone quello che la

ricordo ai colleghi che sull'ordine dei lavori almeno ai rappresentanti dei Gruppi non mi pare che la parola sia stata mai tolta. Oppure abbiamo cambiato il Regolamento anche su questo? Magari non me ne sono accorto e nella notte abbiamo cambiato il Regolamento, e quindi ai rappresentanti dei Gruppi non è più consentito intervenire. Signor Presidente, siccome lei, come me e come gli altri Presidenti

di capire che lei aveva dato la disponibilità a concedere qualche minuto in più. Se questo è diventato un problema, ne prendiamo atto e apriamo un dibattito su tutto il resto - avrei voluto chiedere al ministro Ciriani se sono in arrivo i quattro emendamenti

sta andando avanti, forse sarebbe il caso di consentire ai colleghi di completare l'illustrazione degli articoli e degli emendamenti. Presidente Boccia, sono d'accordo su quello che era stato concordato durante la riunione dei Capigruppo. Le comunico che al Gruppo Partito Democratico sono già stati concessi quattordici minuti in più di quello che era stato stabilito.

possa però essere un elemento di riflessione per tutti su una questione importantissima da riconsiderare in legge di bilancio, cioè il rifinanziamento del fondo Alzheimer, che è stato istituito nel 2021 a seguito di un lunghissimo lavoro cominciato nel 2014 con l'approvazione del Piano nazionale

Siete d'accordo? Tutti siete d'accordo a votarlo per parti separate? I Capigruppo cosa mi dicono? Va bene, votiamolo per parti separate. Io dico semplicemente una cosa: lo votiamo per parti separate sapendo che c'è il parere contrario di relatori, Governo e 5a

sarò telegrafica nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle su questo emendamento, d'accordo con il mio Capogruppo. Chiedo di aggiungere le firme di tutto il Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Siccome questa sarà materia di discussione anche in legge di bilancio, non so se tutti sanno che dal 2014 in Italia abbiamo un Piano nazionale demenze, che non è mai stato finanziato. In Francia hanno previsto nel loro piano 2 miliardi, giusto per far capire la dimensione delle cose. Nella scorsa legislatura abbiamo creato un fondo

vengano ulteriormente spezzettati e destinati ad altro. Se vogliamo fare un'azione unita, tutta l'Assemblea insieme con il Governo, visto che qui lo sollecito, finanziamo il Piano nazionale demenze. È una cosa importante: un milione e mezzo di cittadini sono coinvolti da questa malattia, tre milioni di famiglie nel nostro Paese. Voi capite che 15 milioni in un fondo non danno risposte alla ricerca, ai farmaci e a tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Quindi dichiaro il voto contrario alla lettera *b)* di questo emendamento e favorevole a tutto il resto.

vorrei spiegare a tutti di cosa si tratta. L'articolo 18 conferisce un *bonus* ai lavoratori a *part-time* ciclico verticale, di cui in quest'Aula ho già parlato diverse volte. Sono prevalentemente lavoratori delle

se non sbaglio, questa maggioranza ha detto più volte di essere contraria alla politica dei *bonus*. Vediamo invece che ricorre agli stessi strumenti che tanto ha criticato,

per dare due volte un *bonus* che non serve in ordinaria amministrazione, che noi avevamo proposto durante la pandemia, in una situazione di emergenza, affiancando una soluzione strutturale. Invece voi la soluzione strutturale l'avete cestinata e continuate con la politica dei *bonus*, che avete criticato.

Passiamo alla votazione

Passiamo alla votazione dell'emendamento

Io vorrei trasformare quindi questo emendamento in un ordine del giorno per impegnare il Governo a trovare una soluzione, perché una soluzione va trovata, La cosa che non è accettabile è che su questo tema è un anno che si dica sostanzialmente no. La cosa sta peggiorando, sta degenerando. Il rischio di fallimento delle imprese è reale, lo dichiarano le imprese e le associazioni imprenditoriali,

Presidente, questo emendamento noi lo abbiamo presentato avvalendoci del

rispettato da parte di tutta l'opposizione, che ha consentito al Governo di non strozzare i tempi con una fiducia. Quando si vuole, quindi, come si è visto, è possibile mettere in campo delle azioni che contemperino l'esigenza di convertire i decreti e di assicurare una discussione parlamentare. All'interno di questo *gentlemen's agreement* c'era anche che avremmo voluto, come facciamo in questa circostanza, inserire nel dibattito alcuni temi che poi riprenderemo nella discussione della manovra di bilancio. Questo è uno di quelli, perché noi riteniamo che sia indispensabile riprendere in mano la questione dei cosiddetti cervelli in fuga dall'estero, questione che il Governo ha impropriamente penalizzato attraverso uno strumento fiscale all'interno del disegno di legge di bilancio. Il Governo, in questo momento, dà parere contrario a questo tema. Vogliamo allora dire, con grande tranquillità, ma anche con grande determinazione, che noi non ci fermeremo a questo livello. Il tema del rimpatrio dei cervelli, attraverso il ripristino integrale delle modalità fiscali previste in precedenza, sarà tema che riproporremo all'attenzione della Commissione e all'attenzione dell'Aula,

Presidente, prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto che, come ha ricordato poco fa il senatore Enrico Borghi, arrivano al termine di una settimana molto complessa, caratterizzata da rinvii e ritardi, vorrei dire che questo è l'ultimo miglio per la maggioranza per provare a incidere, attraverso i Gruppi parlamentari, sull'impianto della manovra. Come è noto, infatti, la maggioranza non ha presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio, quindi ha riversato tutte le proprie speranze sul Governo che corregge se stesso. sede perché non abbiamo l'occasione di tornare in Conferenza dei Capigruppo, a meno che lei non ci dia informazioni diverse (ma immagino di no),

i quattro emendamenti del Governo. Ministro Ciriani, ci auguriamo che arrivino nella giornata di oggi, anche se per la verità li aspettavamo ieri. Quello che oggi segnaliamo, presidente Centinaio, è che alla fine di questo provvedimento la maggioranza ha trovato le risorse (diverse centinaia di milioni di euro e il senatore Manca in dichiarazioni di voto

e le demenze; insomma non ha trovato le risorse per gli italiani che soffrono. *(Applausi)*. Allora, signor Presidente, io mi auguro che oggi arrivino gli emendamenti del Governo che correggono il Governo e che forse forse provano a interpretare le speranze vane della maggioranza. Se così non dovesse essere, signor Presidente, nelle ore successive noi chiederemo un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo, perché dovremo rivedere i tempi

all'inizio pensavo fosse fossero divisi per competenze specifiche, perché la manovra è fatta di tre tomi molto pesanti, invece semplicemente ognuno controlla l'altro, perché tre Gruppi parlamentari divisi su tutto devono controllarsi tra di loro. Signor Presidente, ci mettiamo nelle sue sagge mani, nella consapevolezza che la Presidenza vorrà garantire che tutti i Gruppi parlamentari possano vedere rispettate le proprie richieste.

a carte, testi, documenti che stanno girando, come spesso accade, e che rappresenterebbero

Se così fosse, è chiaro che concordo col senatore Boccia, nel senso che va rivisto completamente il calendario delle prossime settimane.

Ho una grande preoccupazione. Mentre alla peggio un decreto scade e si arriva all'ultimo giorno utile per convertirlo, non approvare la legge di bilancio il 31 dicembre significa portare il Paese in esercizio provvisorio. Ho il timore e il sospetto che ci si arriverà per incapacità totale di Governo e maggioranza nel gestire un percorso che, grazie alle opposizioni, è ordinato, ma che non sarà sicuramente grazie alle opposizioni che si porterà a termine.

in molti casi non saranno prese neanche nella legge di bilancio e, quindi, le risposte sui temi della previdenza, della sanità e di tanti altri argomenti che sono contenuti in questo decreto resteranno senza risposte ancora per diversi mesi. mesi. Prima di entrare nel merito, desidero ringraziare il Presidente della Commissione bilancio e i relatori per l'importante lavoro svolto in Commissione e fare due considerazioni. La prima è che il no del Governo alla presentazione di emendamenti alla legge di bilancio ha fatto sì che i membri della maggioranza portassero in questo decreto le loro istanze. Ciò ha snaturato in parte il decreto che, da titolo, doveva affrontare solo le questioni indifferibili per diventare a tutti gli effetti parte della legge di bilancio, ma senza i tempi di discussione e i margini di agibilità che competono alla manovra economica. Appare quindi del tutto evidente che la richiesta di non presentare emendamenti alla più importante legge che ogni anno il Parlamento è chiamato a esaminare sta producendo una distorsione sull'esame dei provvedimenti. L'abbiamo visto plasticamente in questo provvedimento e temo che lo vedremo anche nei provvedimenti economici del nuovo anno. Dall'inizio della legislatura, il Governo ha emanato 47 decreti-legge. Con questa media saranno 200 decreti in cinque anni contro i 146 della XVIII legislatura e i 100 della XVII. poi il costante ricorso alla questione di fiducia: 42 volte nei primi 400 giorni, da parte di una Presidente del Consiglio che oggi fa esattamente quello che criticava ai suoi predecessori quando era all'opposizione. segnalo l'impossibilità nel portare avanti iniziative legislative di origine parlamentare, come se il Parlamento fosse solo il luogo della ratifica burocratica o quello solamente chiamato alle celebrazioni e alle commemorazioni. Mai come ora il Parlamento dovrebbe difendere le sue prerogative, a partire proprio dai colleghi della maggioranza che sono stati privati della possibilità di portare in legge di bilancio le istanze del proprio territorio, i temi in nome dei quali sono entrati in Parlamento. La seconda considerazione è che il provvedimento che oggi votiamo contiene sicuramente alcune misure positive. Tuttavia - come rilevo anche sul proroga termini - la sensazione è che molte di esse non siano in un quadro organico. Si riduce l'IVA sui ritocchi estetici, ma nel frattempo in legge di bilancio si aumenta quella sui beni di prima necessità per l'infanzia; si guarda inermi alle legittime proteste degli operatori sanitari e si cerca - è il caso di dirlo - di indorare la pillola rinviando la fatturazione elettronica per i medici. Si introduce il codice per gli affitti brevi, ma non si fa una riflessione su come le piattaforme digitali hanno stravolto il mercato immobiliare, rendendo le nostre più importanti città un *bed and breakfast* a cielo aperto, con buona pace delle famiglie, degli studenti, dei commercianti e delle piccole imprese, che non riescono più a prendere in affitto un locale o un appartamento. Gli elementi migliori, Presidente, sono negli aiuti alla Toscana, nella proroga dell'assistenza ai profughi ucraini e nell'estensione del fondo di garanzia per il terzo settore. Sempre sul terzo settore, tengo a ringraziare la Commissione per l'approvazione del mio emendamento con cui si estende al 2024 la possibilità per le ONLUS di poter accedere al 5 per mille della dichiarazione dei redditi. Quello che invece ci preoccupa, Presidente, è che tutte le proposte volte a sciogliere i grandi nodi sono state respinte. Penso a quelle per il rafforzamento del trasporto pubblico locale e, soprattutto, per la proroga del mercato tutelato. È ovvio che la libera concorrenza porta beneficio al consumatore. Ma la libera concorrenza si concretizza quando le imprese sono obbligate a competere e quando i cittadini non sono sommersi da pratiche commerciali aggressive o da comunicazioni mendaci. In questo caso si chiama giungla. ARERA ha stimato che il 61 per cento delle persone che hanno accettato un nuovo contratto si è trovato a pagare bollette più salate di prima; solo lo 0,8 ha conosciuto una forte convenienza economica. Per questa ragione, prima di passare al mercato libero, occorreva sminare il campo da tutto quello che ha reso questo mercato un vero e proprio incubo per le famiglie. Era questa la questione che il Governo doveva portare in Europa, come era stato chiesto anche dall'ordine del giorno approvato in Commissione e sottoscritto anche da alcuni membri della maggioranza. Purtroppo, però, così non è stato. Vi limitate a un monitoraggio sui prezzi che ricorda iniziative come il cartello dei prezzi medi della benzina o il carrello della spesa calmierato. Sfido a trovare una sola persona che dica che, dopo queste iniziative, i prezzi dei generi alimentari sono scesi.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, iniziamo con due notizie positive, ringraziando ovviamente anche noi il Presidente della Commissione bilancio e il relatore per aver approvato due emendamenti a cui teniamo molto. Il primo è sul trasporto pubblico locale: una vera rivoluzione, che prende spunto da un disegno di legge presentato nella passata legislatura dalla collega Paita e soprattutto dalla collega Noja. ribalta il modo con il quale vengono dati i finanziamenti al trasporto pubblico locale, nel senso che vengono finanziate le società e le aziende che hanno un piano anche per quanto riguarda il trasporto dei disabili.

le mancanze dello Stato, della macchina pubblica, ad esempio, per tutto ciò che riguarda la gestione dei migranti. È quindi un elemento importante, di grande civiltà. Al netto di queste due buone notizie, l'esito di quello che viene chiamato decreto anticipi - in teoria doveva anticipare parte della manovra e forse consentire alla maggioranza di poter presentare gli emendamenti che in manovra invece non le è stato consentito fare

visione strategica. Cerco di declinare quanto detto in tre esempi. In primo luogo, non sono stati dati pareri favorevoli agli emendamenti che riguardano il mondo dell'agricoltura; mondo che, al netto delle fotografie fatte dai presidenti delle grandi associazioni, in realtà vive un momento di grande difficoltà, perché ha appena subìto dei danni alluvionali non da poco in alcune Regioni importanti per il mondo agricolo; una legge di bilancio un po' avara nei suoi confronti. Ad esempio, non è stata concessa la detrazione Irpef alle aziende agricole, come se le aziende agricole fossero di serie B.

il ministro Musumeci voleva che le assicurazioni dessero il loro assenso a tutte le case dei cittadini italiani per un'assicurazione contro i danni; addirittura nel disegno di legge di bilancio c'è questo per quanto riguarda gli strumenti delle aziende; agli agricoltori, invece, che hanno bisogno dell'assicurazione per eventi calamitosi, questa viene decurtata. È evidente,

a quello che furono gli 80 euro di renziana memoria: sono comunque molti di meno e in molto meno tempo. C'è una certa propensione a cercare delle risorse per le pensioni, ma

Infine, per quanto riguarda il rientro dei cervelli, si tratta di un tema delicato: noi abbiamo ricevuto da parte di molti lavoratori e di molti italiani all'estero una richiesta di revisione totale di quelle norme. quelle norme. Spesso gli italiani non vanno all'estero perché sono felici di andarci, ma perché vedono lì la possibilità di realizzare i propri sogni. Penso in primo luogo alla categoria dei ricercatori, che - non so perché - in Italia non riescono ad avere fortuna se non hanno un certo pedigree e una certa tradizione di famiglia. All'estero, invece, la formazione della scuola italiana, che è ancora una delle migliori, viene apprezzata talmente tanto che sono i nostri ricercatori a essere chiamati a gestire molte ricerche. Ricordiamo che furono i ricercatori italiani a scoprire il Covid: tre ricercatrici donne, per la precisione. Allora, farli rientrare in Italia significa far rientrare persone che abbiamo formato noi fino ai

un comparto che non ha mai avuto grandissime risorse. Signor Ministro, non si preoccupi: abbiamo avuto periodi di magra; poi si è cercato di cercato di correre ai ripari in questi anni e, anche attraverso le risorse del PNRR, si poteva dare una svolta. Invece, si ha una visione che francamente non ci aspettavamo di chiusura, di un ritorno al passato di cui questo Paese non aveva bisogno. Di tutto ha bisogno di questo Paese tranne che di risorse per quanto riguarda la formazione, la cultura e l'integrazione dei giovani nel mondo del lavoro. Allora, come diceva il collega Patton, più che di anticipi si tratta di ritardi: ritardi strutturali per un Paese che di questi ritardi non ha bisogno. Questo Paese ha bisogno di una svolta radicalmente opposta, di risorse e di visioni strategiche perché il mondo sta cambiando e il periodo è difficile: la nostra economia

allora lo 0,7 per cento è una pallida fotografia di quello che fu. Proprio perché è una pallida fotografia, le risorse che ci sono oggi

di una realtà fatta di cittadini che, al netto dei proclami e delle fotografie di rito del Governo, fanno fatica ad arrivare a fine mese. Non c'è nulla

in modo condiviso tra maggioranza e opposizione. Anch'io riconosco al presidente Calandrini una gestione corretta,

erano tutti costosi. Per quanto riguarda gli emendamenti delle opposizioni, si è chiuso su tutte le richieste che si facevano; mentre dall'altro lato

abbiamo cercato di affrontare un metodo e di rispettarlo, dopodiché la maggioranza non l'ha rispettato per niente. Quanto al merito, si è detto di no a una serie di temi che ho cercato di illustrare anche durante la discussione e la presentazione degli emendamenti,

Ad esempio, non si è affrontato un tema fondamentale. Noi siamo in una situazione in cui in tutto il Paese è emersa con forza,

stanno intaccando i risparmi, nel nostro Paese, per poter andare avanti. È chiaro che, a questo punto, si spingono i figli a frequentare università

Se il buongiorno si vede dal mattino e se questo era il decreto anticipi della finanziaria, cosa posso aspettarmi dalla finanziaria? Questo mi pare il dato fondamentale. Posso andare avanti: pensiamo a tutta la fragilità.

ci sono le guerre e il clima cambia. Pensiamo alla questione della transizione ecologica, a rendere il nostro Paese più autonomo nella produzione. Se si deve fare questo, bisogna investire sul nuovo,

anche stamattina in Commissione. È chiaro che, se il Governo arriva con 15 emendamenti, e quindi emenda sé stesso - a parte il fatto che aveva

un'altra volta questa impostazione e poi alla fine avere due dita negli occhi. Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, vorrei iniziare questo intervento innanzitutto in controtendenza rispetto a quanto detto dal senatore Magni, ringraziando il Presidente della Commissione bilancio, i relatori e il Governo per aver individuato un metodo di lavoro condiviso. In Commissione ci si è confrontati nel merito - come ricorderà Borghi - anche con le opposizioni e il testo del decreto è stato integrato con parecchie norme utili e funzionali alla *ratio* complessiva del provvedimento. È un decreto fondamentale per i numeri del bilancio dello Stato del 2023 e lo è ancora per i riflessi che si hanno e si avranno sul 2024. A parlare sono soprattutto le poste economiche, che utilizzano integralmente i 18,2 miliardi di maggiore indebitamento deliberato dalle due Camere - come ricorderete - l'11 ottobre del 2023. In particolare, si tratta di 17,5 miliardi di maggiori spese e 700 milioni di minori tasse. Ma sono numeri che certamente si riverberano anche sul bilancio 2024, visto che vengono anticipate al 2023 molte poste del prossimo anno. L'impostazione è quella di un decreto molto razionale e soprattutto equilibrato, proprio come la legge di bilancio 2024 che stiamo esaminando in Commissione bilancio. Anche i numeri sul 2024 vedono un sostanziale bilanciamento tra entrate per 2,389 miliardi e spese per 2,407 miliardi di euro. La novità di questo Governo e della maggioranza sta proprio nel misurare l'equità delle misure e le risorse per farvi fronte. Si tratta di norme di buon senso, che sono dirette a quella ampia platea di persone che ha sofferto di più negli ultimi anni di congiuntura negativa, salvaguardandone il reddito. Viene aumentato il potere di acquisto dei pensionati, con quasi 1,5 miliardi di euro, anticipando di un mese, al 1° dicembre 2023, la decorrenza della perequazione automatica delle pensioni. La perequazione è a valere sui ratei dei trattamenti pensionistici di tutto il 2023. Vi è poi il tema degli statali che rinnovano i contratti, per i quali viene prevista una indennità di vacanza contrattuale che copre il periodo di dicembre 2023. Due miliardi e mezzo vengono dedicati al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi dei lavoratori autonomi con dichiarazione sotto i 170.000 euro. Questo anticipo può essere dilazionato tra gennaio e maggio in cinque rate mensili. Viene introdotto un contributo di solidarietà, stimato in 450 milioni di euro per il 2024, a carico delle imprese del settore energia che in questo periodo hanno fatto i maggior profitti. Poi c'è un capitolo di disposizioni dedicato a perequare il trattamento degli enti territoriali. In particolare, vengono dati 300 milioni di euro alla Regione Sicilia per provvedere al fabbisogno sanitario regionale del 2023; 25 milioni di riduzione del concorso alla finanza pubblica al Trentino-Alto Adige; 40 milioni vanno a ciascuna Provincia autonoma di Trento e di Bolzano a titolo di compartecipazione del gettito delle accise petrolifere; a Bolzano vanno anche 24 milioni di compensazione degli oneri previsti dalla convenzione con la Rai. milioni vanno alla Regione Molise come contributo vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione. Viene rifinanziato con 500 milioni per il 2023 il fondo per il trasporto pubblico locale; 35 milioni vanno al cosiddetto bonus trasporti per coprire il costo dell'acquisto di abbonamenti al È previsto anche un emendamento, introdotto in Commissione bilancio, per il differimento dei termini relativi agli adempimenti contributivi e previdenziali delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato colpite dagli eventi calamitosi del 2 novembre. Contrariamente a quello che è stato detto, non siamo stati insensibili al trovare le soluzioni per le popolazioni che hanno subito una tale sventura. Poi c'è il capitolo infrastrutture. Per gli alloggi e le residenze universitarie vengono stanziati 96 milioni come cofinanziamento del *target* previsto dal PNRR per lo stesso scopo. Per coprire i fabbisogni di cassa del 2023 di RFI (Rete ferroviaria italiana), sia per nuove opere che per la produzione straordinaria, viene stanziato un miliardo di euro. Inoltre, ci sono i contributi agli investimenti. La nuova Sabatini a favore delle piccole imprese viene rifinanziata con 50 milioni. Ai programmi della difesa e di elevato contenuto tecnologico in campo aeronautico vanno 326 milioni. Vi sono misure a sostegno delle imprese esportatrici, attraverso una norma inserita in Commissione bilancio. Sempre in Commissione bilancio, è stata aggiunta una norma che rilancia il fondo di garanzia per le PMI. Diversi contributi economici vengono stanziati in ambito dello sport,

Infine, vengono incrementate di 15 miliardi, portati a 18,2 miliardi per il 2023, le risorse per l'attuazione del cosiddetto superbonus 110. Ma nel bilancio dello Stato dei prossimi anni, la cessione dei crediti edilizi peserà ancora per circa 23 miliardi ogni anno, con strascichi finora quantificati in 135 miliardi. Un sostegno al settore delle costruzioni e dell'edilizia verrà certamente dai cantieri del PNRR. Con una modifica introdotta in Commissione bilancio, viene ulteriormente rafforzata la capacità amministrativa sia della pubblica amministrazione che dei soggetti attuatori. Per quanto riguarda le ristrutturazioni, che rappresentano la metà del valore della produzione del settore, che è di circa 300 miliardi di euro, il sistema degli incentivi va ricondotto a razionalità e sostenibilità. È quello che sta facendo questo Governo, che è consapevole dell'importanza strategica del comparto edilizia sull'economia nazionale. Concludo ribadendo un plauso al lavoro fatto in Commissione, un lavoro di squadra, in cui i senatori di Forza Italia hanno giocato un ruolo importante e soprattutto determinante, che ha portato a un provvedimento molto concreto. Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia.

Ovviamente, non possiamo che essere contenti della proroga dello *smart working* nel settore privato; come ho detto già ieri, sarebbe stato bello avere tempi più lunghi, dato che è stato concesso solo fino al 31 marzo, e mi auguro che sappiate che c'è il problema del settore pubblico, per cui questa proroga non è ancora stata concessa e auspico che arrivi. Non posso che essere più che soddisfatta di quello che è accaduto poche ore fa in quest'Aula, quando tutti i Gruppi parlamentari hanno messo la firma su un mio ordine del giorno volto a istituire un fondo per l'acquisizione di macchine come quelle per la perfusione che si utilizzano per i trapianti. È stato certamente un momento di unità e di propositività di questo Parlamento; esulteremo di più quando questo

si parla di un decreto-legge a tutela del lavoro per le esigenze indifferibili, che dovrebbe promuovere la crescita e azioni

non si capisce da che parte volete andare o, meglio, si capisce benissimo: come al solito, state legiferando in maniera da avvantaggiare pochi, che erano già beneficiari di numerosi vantaggi e in una posizione economica eccellente, e continuate a svantaggiare le classi già sfavorite della popolazione; ad esempio, nel provvedimento in discussione anticipate il taglio dei fondi per la disabilità e avete respinto tutti gli emendamenti, come abbiamo visto poco fa, che andavano a rifinanziare una serie di fondi per la non autosufficienza, la disabilità o l'Alzheimer. *(Applausi)*. La quantità di tempo che ci siamo presi in quest'Aula per illustrare gli emendamenti e discuterli fa ben capire quanto siate lontani dalla realtà del nostro Paese e ci state portando in una direzione che che non è quella che serve all'Italia. Sono più le cose che non ci sono nel decreto-legge che quelle che ci sono; a parte la fortuna che non ci sia, come ho detto ieri, l'emendamento per consentire ai condannati di entrare di nuovo nei Comuni

che stanno affrontando il caro mutui; non volete aiutare il Paese a fare una vera transizione energetica, non fate niente per il credito d'imposta per chi acquista impianti da fonti di energia rinnovabili e non volete abolire i sussidi ambientalmente dannosi. Mi domando cos'è che volete fare, a parte aiutare le banche e gli altri che fanno extraprofitti. *(Applausi)*. Vi siete insediati dicendo che eravate il Governo del lasciar fare a chi vuole fare, neanche questo state mantenendo: state affossando persino le imprese che ci hanno aiutato ad alzare il PIL subito dopo la pandemia, i cosiddetti esodati del superbonus, piccole imprese italiane che avevano in pancia tantissimi crediti del superbonus, strumento che raccontate ovviamente malissimo, accusandolo di essere colpevole di un buco di bilancio che però nei conti pubblici non esiste. Ribadisco ancora una volta non c'è nessun documento che attesti che esiste il buco di bilancio che andate raccontando voi, mentre ci sono tantissimi documenti che attestano quanto la misura abbia spinto il PIL, abbia fatto aumentare l'occupazione

Voi invece, nel cosiddetto decreto sulla circolazione dei crediti d'imposta, la circolazione dei crediti l'avete cancellata. Adesso andate raccontando che le imprese sono in difficoltà per colpa della nostra norma, mentre in realtà sono in difficoltà perché non hanno più potuto cedere i crediti perché voi glielo avete impedito.

che per l'anno prossimo il PIL del Paese sarebbe cresciuto dell'1,2 per cento, ma adesso le stime sono già allo 0,7 per cento. Questo differenziale è quello che vi avrebbe permesso di decantare una fantomatica riduzione del rapporto debito-PIL e che invece, a causa delle mancate misure per la crescita del Paese che voi non avete adottato, crescerà. Il buco di bilancio lo avete fatto voi e lo vedremo l'anno prossimo. *(Applausi)*. Non avete neanche prorogato le misure a favore dei territori colpiti dal sisma e dall'alluvione. Vi accanite, cioè, contro chi è in difficoltà, difficoltà, come gli studenti fuori sede, perché la Ministra va a parlare di alloggi, di residenze e di misure che possano favorirli, ma poi nella pratica tutte le proposte che vi vengono fatte in questa direzione naturalmente le bocciate. le nostre imprese chiedono un quadro normativo chiaro e duraturo per poter programmare e fare investimenti e aumentare l'occupazione, ma voi non lo fate. Le misure più utilizzate dalle imprese per l'innovazione tecnologica e per guardare al futuro, come Innovazione 4.0, le avete trasformate rendendole inutili, non le prorogate e non accogliete neanche gli emendamenti che vi suggeriscono cosa fare quando non siete capaci di capirlo da soli. Niente, assolutamente niente. La stessa cosa accade con la Strada dei parchi, com'è stato detto prima: avete tradito tutte le promesse fatte, avete tradito i sindaci e avete tradito i pendolari che percorrono quella strada ogni giorno a tariffe altissime. Tante promesse in fase pre-elettorale, ma anche subito dopo, e poi nei fatti andate in direzione completamente opposta. Vi siete dipinti come il Governo pronto ad affrontare le sfide e la guida del Paese, ma a noi sembra che ci stiate guidando direttamente dentro il baratro della recessione. La vostra manovra doveva essere seria, prudente e responsabile, ma siete responsabili solo nei confronti di chi ha già tanto e invece siete totalmente irresponsabili nei confronti dei cittadini di questo Paese. Per questi motivi, il nostro

il conguaglio dell'incremento pensionistico che questo Governo ha riconosciuto a tutti i pensionati (ricordo che stiamo parlando di 16 milioni di persone). Il fatto di far avere questo incremento a dicembre, invece che l'anno prossimo, secondo me è stata una cosa gradita da parte di molti pensionati, come penso che chiunque abbia potuto verificare. Stiamo parlando però di 1,4 miliardi di euro.

Vorrei ricordare che sempre in questo decreto-legge ci sono altri due miliardi per l'incremento e l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, tutte misure giuste; non stiamo regalando niente a nessuno, questo dev'essere chiaro. I pensionati hanno diritto alla loro rivalutazione e i dipendenti pubblici hanno diritto al loro contratto, questo dev'essere chiaro. In passato le pensioni non sono mai state rivalutate (quantomeno negli ultimi dieci anni), anche quando si era in presenza di incrementi molto più piccoli dell'inflazione, anzi, in certi casi impercettibili;

parte tutto. Almeno si fa un po' di chiarezza sulle pensioni perché, in modo assolutamente strumentale, tante volte dall'opposizione ho sentito dire che si fa cassa sui pensionati perché magari a chi aveva 10.000 euro di pensione non è stato dato l'aumento di 1.000 euro al mese.

su tutte le pensioni di 16 milioni di cittadini. Sono state cifre molto importanti, che hanno pesato sul bilancio. Oggettivamente però questo provvedimento arriva a 16 milioni di cittadini. Il superbonus è arrivato a

È diritto di un lavoratore avere il contratto aggiornato perché anche per il lavoratore, come per il pensionato, se il contratto non viene aggiornato, in presenza di inflazione, c'è una riduzione reale dello stipendio. stipendio. Stiamo parlando in ogni caso di diritti, ma anche in questo caso, se c'è una vacanza contrattuale, è perché da anni non sono stati rinnovati. Anche sul fatto che ci fosse un'enorme inerzia nel rinnovo dei contratti stiamo vedendo un intervento obiettivi che erano attesi in certi casi da anni e che spero si raggiungano in modo definitivo. D'altra parte, nel disegno di legge di bilancio ci sono le risorse, specialmente per alcune categorie più numerose, in modo tale da non avere un'indennità di vacanza contrattuale, ma l'effettivo rinnovo del contratto.

mi sembra che non sia mai stato ricordato abbastanza il colpo di mano del Governo precedente, nello specifico probabilmente del Presidente del medesimo Governo, che era il migliore e non falliva mai (però in questo caso forse un po' gli era scappata la "miglioranza"), il quale aveva espropriato, probabilmente in maniera illegittima, a giudicare da quanto dicono i tribunali, un'autostrada a un concessionario,

5 miliardi significa non poter rinnovare i contratti di cui sopra, significa non poter pagare le pensioni di cui sopra e così via. Quindi, se il Governo - penso sia stato riconosciuto più o meno da tutti - è riuscito finalmente a trovare

Sempre fra i buchi che si cerca di coprire, non si è parlato per niente di trasporto pubblico locale. In questo provvedimento ci sono 500 milioni per il trasporto pubblico locale in certi casi, con i soldi messi da questo Governo, tanti sindaci di sinistra fanno la ruota come i pavoni, dicendo di essere bravi. Sono bravi, ma probabilmente perché c'è un Governo che li supporta, com'è giusto che sia, perché garantire il diritto di spostarsi in modo efficace ed efficiente ai cittadini non è né di destra, né di sinistra *(Applausi)*, ma questo Governo cerca di andare incontro esattamente a queste esigenze. Mi auguro che venga riconosciuto o quantomeno che ne venga preso Seppure sarebbe stato piacevole, utile e doveroso fare di più subito, c'è anche un inizio di intervento nei confronti delle aree alluvionate della Toscana. Magari uno non alluvionate della Toscana. Magari uno non ci pensa, ma non è questo l'intervento a favore delle aree alluvionate; serve esclusivamente per evitare un'ingiustizia terribile, vale a dire che chi in quel momento aveva la casa

contingente, com'è giusto che sia in un decreto-legge in cui bisogna affrontare le questioni urgenti: bisogna evitare la beffa che qualcuno, magari evacuato o scappato da casa, perché era scattata l'evacuazione per pericolo di inondazione, debba addirittura prendere una multa per quello che è successo. Credo quindi che ci siano aspetti molto positivi in questo decreto-legge e sono contento che alla fine l'abbiamo esaminato con un certo grado di accordo, più o meno fra tutti. Un'ultima cosa, prima di chiudere: vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo presenti in Aula che quando il livello di "parere-contrarismo", per così dire, comincia a salire oltre un certo livello, forse una qualche riflessione va fatta.

che, con una certa leggerezza, ricevono parere contrario dal Governo o dai Ministeri (non si riesce mai neanche a capire bene quale sia l'origine di questi pareri contrari)

Quindi la prossima volta, se arriva qualche altissima parte del nostro ordinamento repubblicano a dire che forse un determinato emendamento non va bene, noi lo approviamo e poi quella lo stralcia, perché la faccia davanti agli elettori la mettiamo noi, non lei.

decreto-legge anticipi anticipa purtroppo una manovra senza respiro, che risulta espansiva solo nei dettagli delle regole di finanza pubblica perfino nel confermare misure già in essere, come il cuneo contributivo, che noi abbiamo condiviso, ma che voi non siete stati in grado di rendere strutturale nell'interesse generale del lavoro e delle imprese. È una manovra inefficace per rilanciare la crescita. C'è un grande assente nel dibattito di oggi. Il fatto che il Governo e i relatori abbiano rinunciato alla replica in questa sede conferma l'assenza di idee e di progetti *(Applausi)* e la difficoltà a rappresentare un'idea dello sviluppo economico e sociale di questo Paese. È una manovra inefficace perché c'è un grande assente, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che resta l'unica leva per favorire investimenti pubblici e privati in una stagione nella quale le imprese e l'economia non crescono. Eppure, non c'è alcun collegamento tra la politica economica di questo Governo e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è il pilastro fondamentale per intercettare i cambiamenti in campo energetico, sociale e digitale per innovare questo Paese e garantirgli un futuro positivo per una nuova crescita economica. L'Europa e l'Italia non possono essere un mercato; sono un luogo produttivo, di crescita, di lavoro e di opportunità. Voi rinunciate a tutto questo e ci presentate una manovra che attacca al cuore il pilastro dei diritti.

quando in realtà sono investimenti fondamentali per un'idea di sviluppo economico, di società e di riduzione delle disuguaglianze? *(Applausi).* Di fronte a noi, ovunque ci giriamo, c'è la grande questione educativa. Considerare l'istruzione e la salute come un costo e non come un investimento rappresenta per me il fallimento delle vostre politiche di Governo, sulle quali noi abbiamo dimostrato di avere un'idea e una proposta alternativa di società, perché i nostri valori sono incompatibili con i vostri. Presentate una manovra in *deficit* di 15,7 miliardi, ma sia chiaro - lo dico ai colleghi di maggioranza - che non c'è solo improvvisazione e propaganda. Abbiamo visto in questo dibattito, in fase di conversione del decreto-legge anticipi, tanta improvvisazione e tantissima propaganda. È evidente che abbiate costruito una manovra in cui il decreto-legge anticipi anticipa in qualche modo i saldi di finanza pubblica dentro i quali dovrete muovermi per questa manovra. sono solo improvvisazione e propaganda. Per noi, il vostro è uno schema vecchio, tipico di tutti i Governi di destra, e lo voglio riassumere in questo modo: nessuna politica industriale; pensate che basti il mercato, senza lo Stato, per agganciare i fattori del cambiamento. In realtà, è il mercato che ha bisogno di più Stato, perché la transizione energetica e digitale richiede un progetto per lo sviluppo; richiede un piano industriale che voi non avete e che negate; richiede di abbracciare la questione dei cambiamenti climatici come un'opportunità, non come un problema. Invece voi li negate anziché valorizzare e regolamentare le comunità energetiche, parlate di nucleare di terza generazione. Voi avete la propaganda perché il vostro obiettivo in questa manovra non è il Paese

quale sarà l'esito di questa tornata elettorale, ma lo fate purtroppo dimenticando che avete avuto la responsabilità di governare il nostro Paese e che lo state facendo senza un'idea di futuro, anzi mangiando futuro. futuro. In questo momento avremmo bisogno di discutere delle riforme e di affrontare, ad esempio sul terreno della salute e dell'istruzione, perfino una riclassificazione della spesa pubblica. Dovreste andare a Bruxelles a discutere del Patto di stabilità e della riclassificazione con Eurostat, pensando che una parte fondamentale della salute non può essere contabilizzata per cassa, quando la ricerca e l'innovazione hanno portato medicinali, farmaci e soprattutto opportunità per prevenire, anziché curare, che rappresentano il più grande e importante investimento per questo Paese. Rinunciate al terreno delle riforme e rinunciate dunque a confrontarvi su un'idea di società e di comunità. Ora, lo dico, questo decreto anticipi è anche l'anticipo del vostro fallimento. *(Applausi)*. Per me è l'anticipo della rinuncia a dare attuazione al programma di mandato. È facile presentarsi agli elettori con più pensioni per tutti

Chi è che ha bisogno della benzina? Spesso è il lavoratore, spesso sono le persone più deboli, che si recano sul luogo di lavoro. Un conto è la propaganda, un altro conto è l'esercizio del Governo. Lo dico perché il vostro programma di mandato prevedeva e prevede meno tasse per tutti. Ecco, riemergono in questa sede, attraverso un emendamento parlamentare, per cui il lupo perde il pelo, ma non il vizio, operazioni che si devono chiamare con il loro nome. Quando un parlamentare in quest'Aula presenta un emendamento, con il consenso del Governo, per intervenire sulla rottamazione-*quater*, a rate già scadute, per noi questo si chiama condono.

sapete perfettamente chi non ha pagato, dovete dare una mano a coloro che non hanno rispettato un patto fiscale tra lo Stato e il contribuente. *(Applausi)*. Questo per noi è il vizio: condoni, anziché un lavoro necessario sul recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale. Io continuo a pensare che chiunque governerà questo Paese debba lavorare per contrastare l'evasione fiscale, non per ampliarla. Allora mi chiedo: come fate a guardare negli occhi i lavoratori e i giovani ai quali avete detto no al salario minimo, quando contemporaneamente lavorate per favorire l'evasione e aiutare l'elusione fiscale? Come fate a pensare e solo ad ipotizzare ciò? Che idea di società avete? Un'idea di società nella quale riducete l'IVA per le attività di chirurgia estetica e per gli integratori alimentari e poi l'aumentate per

Presidente, ringrazio il presidente Calandrini per aver consentito, per lo meno in Commissione bilancio, un confronto evidente e utile. In questo modo, abbiamo evidenziato le nostre proposte, perché, di fronte ai vostri tagli sul pilastro della previdenza, noi rispondiamo con la reintroduzione di Opzione donna e delle misure sociali *(Applausi)*, perché è inaccettabile in questo Paese parlare di politiche di genere e colpire l'uscita dal mondo del lavoro delle donne. È inaccettabile. Non sono politiche di genere, le vostre sono scelte per lasciare da sole le persone più deboli, più fragili. Sono scelte per aumentare le disuguaglianze, perché nella solitudine, cioè in un mercato che da solo fa da sé, si ampliano le disuguaglianze, non ci sarà crescita economica, dovrete ricorrere al taglio dei servizi essenziali ai cittadini dei vostri tagli lineari, quando vi accorgerete che la sostenibilità del debito non c'è senza crescita, dovrete mettere mano al taglio lineare sui servizi, che significa ampliare delle disuguaglianze, lasciare da sole le persone che non ce la fanno, costruire un'idea di società senza coesione e senza comunità. Voi rinunciate al futuro del Paese, in questo modo. Ecco perché avete un'idea sbagliata. Noi abbiamo tentato di produrre in questa sede un'idea di Paese e di società alternativa.

aiutare l'elusione e l'evasione fiscale, pensando che l'unico obiettivo sia capitalizzare le banche, e di non aiutare il lavoro, non alzare i salari e non garantire l'accesso al lavoro in maniera degna ed equa? Poi ci si lamenta che i nostri giovani scelgano una strada per andare fuori dal nostro Paese. Certo, se sono costretti ad entrare a 5 euro l'ora nel mercato del lavoro, perché voi dite di no ai 9 euro del salario minimo, ci sarà una ragione. Avete un'altra idea, corporativa: per voi vengono prima i consulenti del lavoro rispetto ai lavoratori, alle persone, alle imprese e all'idea di società e di sviluppo economico di questo Paese. In conclusione, queste sono le ragioni per le quali le nostre proposte sono incompatibili con le vostre priorità e ne siamo orgogliosamente fieri, perché abbiamo un'idea di società e di Paese alternativa. Voi state sbagliando, ve lo diciamo ora per allora. Non avete una visione lunga. State perfino tradendo il vostro programma di mandato e state dicendo al vostro elettorato che è molto facile promettere, ma poi, purtroppo, la vostra identità e i vostri valori vi portano a favorire un'idea corporativa della società e a demolire la giustizia, l'equità, la solidarietà e la necessità che abbiamo di costruire crescita e sviluppo economico. *(Applausi)*. Per questo voteremo contro il provvedimento

Avete fatto una conversione del decreto anticipi utilizzando circa 800 milioni di euro. Ora fate in fretta, prima che inizi la discussione del disegno di legge di bilancio, a reperire le risorse per gli affitti e a individuare le risorse per contrastare i tagli che avete fatto sulle disabilità, perché noi su questo non arretreremo. Abbiamo bisogno di risorse aggiuntive di risorse aggiuntive per stimolare una ripresa di valori fondamentali per aiutare i giovani, per aiutare le donne e per aiutare un'idea di società alternativa alla vostra. Voteremo convintamente contro.

*(Applausi)*. Vorrei ringraziare ovviamente i relatori, tra cui la nostra senatrice Nocco, il relatore Borghi e il relatore Damiani, vorrei ringraziare tutti i senatori che si sono impegnati nel varare questo disegno di legge così importante. Prima di trattare però di temi economici, credo che sia sempre utile soffermarci un secondo sulla fase congiunturale, storica ed economica che stiamo tutti vivendo, cari senatori. Io ricorderei a tutti noi, che pensavamo che non spirasse più quel terribile vento pandemico, che invece ha cominciato a spirare quello di due guerre ai confini, alle porte dell'Europa. Quindi, indubbiamente viviamo una fase piuttosto complessa. C'è un detto detto che dice: io non auguro a mio figlio di vivere in tempi storici interessanti. Indubbiamente, noi oggi viviamo in tempi storici di interesse. storici di interesse. Quante e quali sono le trasformazioni che stiamo vivendo? Proprio oggi, per esempio, qualcuno richiamava i rapporti con l'Unione europea. In Commissione, abbiamo varato un'importante risoluzione, sia alla Camera che al Senato, in merito alla *governance* europea. Abbiamo chiesto, con quell'atto che è stato approvato stamattina, di andare a rivedere il rapporto *deficit*-PIL del 3 per cento e il rapporto debito-PIL del 60 per cento. Sappiamo e siamo tutti coscienti di quanto sarebbe incredibilmente difficile garantire quella crescita che oggi occorre a tutta l'area euro, se se quei parametri rimanessero in vigore, a prescindere da quelli che siano i regolamenti che verranno applicati dalla Commissione europea. adesso *in medias res*. Io ho avuto l'onore e l'onere di svolgere questa dichiarazione di voto per il Gruppo Fratelli d'Italia.

di anticipo della decorrenza della perequazione automatica per le pensioni a decorrere su tutti i ratei pensionistici del 2023. E questo perché vogliamo sostenere i nostri pensionati.

la possibilità di avere i *fringe benefit* rivalutati, che li portano a quasi una tredicesima in più rispetto a quella che sarebbe stata prevista. Richiamo anche quei 2,5 miliardi dedicati al rinvio della seconda rata dell'anticipo delle imposte dei redditi per tutti coloro che abbiano redditi sotto i 170.000 euro. Noi riteniamo che bisogna sostenere, supportare quello che è un ceto medio - senatori - che ha sofferto molto e che oggi noi riteniamo di andare a sostenere. Qualcuno prima stava richiamando il tema della Toscana. Toscana. È vero che la Toscana ha sofferto ed è per questo che noi abbiamo previsto 50 milioni per le emergenze nazionali e per il fondo a sostegno anche delle imprese esportatrici della Regione Toscana colpite dai recenti eventi alluvionali, con ristori sotto forma di contributo a fondo perduto, attingendo alle giacenze del fondo SIMEST. *Ad adiuvandum,* sempre per chi si preoccupava per la questione della Toscana, della quale anche noi ci siamo preoccupati, la Commissione ha approvato il differimento dei termini per gli adempimenti contributivi e previdenziali di tutta la Regione, colpita appunto dalle alluvioni di novembre. Vogliamo continuare a parlare dell'impresa? Vogliamo trattare del tema del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese? Certo, è un provvedimento composito, perché l'intendimento è partire dal generale, ma anche andare a toccare nel particolare la carne viva delle esigenze, delle varie realtà. E allora come non richiamare, per esempio, il tema del trasporto pubblico? Ho sentito che qualcuno lo ha fatto, con il rifinanziamento di 500 milioni per il 2023 e 35 milioni per il *bonus* trasporti. il contributo di solidarietà, che è stato previsto a carico delle imprese del settore delle energie. Altro che abbandono delle categorie dei vulnerabili da parte nostra. il 5 per mille per le ONLUS e la relativa proroga. Noi riteniamo che, in virtù del principio di sussidiarietà, ci sia quella valenza sociale che deve essere sempre da noi adeguatamente sostenuta. La formazione è uno dei temi che mi sta maggiormente a cuore e anche in questo caso andiamo a sostenere la libertà di scelta educativa con i 50 milioni di euro previsti per le scuole paritarie. Qualcuno prima dagli scranni della minoranza si preoccupava dell'edilizia universitaria. Non lo fate, perché noi prevediamo 96 milioni di euro per gli alloggi e le residenze universitarie. un altro aspetto oltre ai sostegni, alle agevolazioni in ambito agricolo, oltre al fatto che continuiamo a dedicare attenzione a quell'ambito per noi fondamentale (*mens sana in corpore sano)* e, quindi, al sostegno adeguato allo sport.

Anche sul superbonus io stessa, in momenti di confronto in seno alla Commissione, avevo chiesto determinati interventi e spero ancora

la sostanza sia chiara a tutti. Ci apprestiamo a varare una manovra di bilancio complessa e, pur tuttavia, manteniamo sempre alta l'attenzione verso le singole esigenze che ci vengono manifestate. Il sommo poeta diceva: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta». Anche oggi la nave è in gran tempesta, ma ringraziando il cielo abbiamo il vantaggio di avere un nocchiere che sa tenere la barra dritta in nome del popolo italiano.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

Signor Presidente, quando penso a Mario Roggero, di professione gioielliere, a tutto quello che gli è accaduto e ha dovuto subire - e non mi riferisco solo agli ultimi avvenimenti, ma a tutta la sua esperienza da commerciante, serio, scrupoloso, vittima di due feroci rapine, una nel 2015 e l'altra nel 2021 - con le drammatiche conseguenze che ben conosciamo, penso a un uomo, a un padre di famiglia, a un lavoratore che più volte ha visto la sua vita e quella dei suoi familiari in pericolo di morte. il suo patrimonio, i soldi raccolti con sudore, con il lavoro suo e della sua famiglia volatilizzarsi in un attimo, strappati via da gente che, a differenza sua, ha scelto la strada del crimine. Ma non basta: possiamo solo immaginare come possa essere trovarsi davanti a un'arma che minaccia me e, ancor peggio, mia moglie e le mie figlie. Ho letto le parole scritte dalla figlia di Mario e mi permetto di citare un passaggio del suo lungo *post*:

Senatrice, la parola «vergogna» la usi a casa sua. Posso chiederle gentilmente di uscire dall'Aula? Quando interviene lei nessuno interviene e nessuno dice niente, almeno quando presiedo io. «In quell'occasione mia sorella maggiore Laura aveva colto in negozio i due malviventi, camuffati da clienti. Mio papà, all'età di 65 anni, era stato picchiato selvaggiamente, ricevendo un pugno in faccia così forte da spaccargli il naso. In una frazione di secondo è affiorato nella mia mente il racconto di Laura, che era stata minacciata con una pistola puntata alla testa, chiusa in bagno e immobilizzata con delle fascette ai polsi. Mi aveva raccontato che aveva chiesto loro in lacrime di non sparare perché aveva due figli a casa. E di nuovo, a distanza di alcuni anni, ecco un'altra aggressione alla mia famiglia». Ricordi che definirei brutali, che mettono i brividi e di fronte ai quali, come rappresentante delle istituzioni, non posso che farmi delle domande. Cosa avremmo potuto e cosa dobbiamo fare noi più e meglio di quanto non sia stato fatto per evitare che simili tragedie accadano? Quali sono le nostre responsabilità nei confronti della famiglia Roggero? Avremmo potuto evitare che il signor Mario fosse costretto a difendere con un'arma la sua famiglia e oggi a rispondere delle sue azioni con una pena sproporzionata. Ancora, cosa avrei fatto io al suo posto? posto? Lo dico qui: aderisco e invito anche altri ad aderire, senza se e senza ma, alla raccolta fondi promossa dalla famiglia Roggero per aiutare Mario e i suoi familiari a sostenere le enormi spese che devono affrontare. Anche questo merita una riflessione, Presidente: per aver difeso il suo lavoro, i suoi sacrifici e soprattutto la sua famiglia, Mario dovrà versare enormi somme di denaro a chi voleva portargli via i soldi e minacciava e malmenava sua moglie e le sue figlie. Personalmente, mi impegnerò e sarò sempre al fianco dei tanti Mario che purtroppo spesso nel nostro Paese si trovano ad affrontare situazioni magari non drammatiche come questa, ma ugualmente dolorose e umilianti. Da quest'Aula, signor Presidente, deve partire un abbraccio forte alla famiglia Roggero, a papà Mario, alla moglie e alle figlie, persone vere che vengono dalla nostra terra, dal Piemonte, dalla Provincia di Cuneo, una terra che tanto dà e mai chiede nulla in cambio. Siamo con voi, Mario, ogni giorno e per sempre. Grazie, Presidente,

Grazie,